dobbiamo ricordare. Dobbiamo ricordare e rendere omaggio alle vittime del criminale disegno nazista di sterminio degli ebrei. Dobbiamo ricordare gli orrendi episodi che si sono verificati anche qui da noi. Bene ha fatto il Presidente della Repubblica, la scorsa settimana, a partecipare a Milano alla presentazione del «Memoriale della *Shoah*»: il binario 21 della stazione centrale come luogo della memoria, quel binario, impiegato negli anni 1943-1944 per la deportazione di ebrei nei campi di sterminio. Su quel binario 21 più di 8.000 ebrei furono stipati nei vagoni, poi piombati prima di farli partire per Auschwitz: pochi, pochissimi ritornarono. Simbolo quindi di barbarie e di vergogna. Dobbiamo non dimenticare, per evitare che si ripetano simili atrocità e anche per prendere la forza per debellare barbarie e genocidi che ancora si verificano. Dobbiamo non dimenticare l'immenso dolore delle persone e delle famiglie coinvolte, l'immenso dolore che tutti devono provare per una tragedia della storia dell'umanità. Un dovere morale, quello di ricordare quegli orrori che hanno negato l'essenza stessa dell'uomo. Per questo voglio anche ricordare un fatto tragico e raccapricciante, forse tra i più disumani; un fatto che ha come sventurati protagonisti venti bambini ebrei, tra i tanti provenienti da diverse località dell'Europa, che, nel 1944, furono trasportati nei *lager* di Auschwitz-Birkenhau. Alla macchina della morte servivano giovani cavie per effettuare assurdi esperimenti sulla tubercolosi. Con un inganno, per non diffondere il panico, Mengele procurò i bambini, dicendo: «Chi vuole vedere la mamma, faccia un passo avanti». Venti bambini furono sottoposti ad esperimenti inutili e a sofferenze disumane. Dopo mesi, Mengele e i suoi criminali colleghi decisero di sopprimerli. Li fecero trasferire alla scuola di Bullenhuser Damm e poi impiccare. Quei corpicini, con i segni della sofferenza, furono poi bruciati per non lasciare tracce; bambini di questa nostra Europa, tra i quali anche Sergio De Simone di Napoli. Allora, venti rose bianche per ricordare; venti rose bianche - dicevo in una precedente occasione - messe a dimora nei giardini di ogni Comune d'Italia per ricordare Sergio De Simone e i suoi piccoli, sventurati compagni. Venti rose bianche anche per sperare, come sperava Anna Frank che scriveva nel suo diario: sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure, partecipo al dolore di milioni di uomini, eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità». È quello di cui ancora oggi abbiamo bisogno. Per questo dobbiamo ricordare e con impegno operare. *(Applausi dei

la quale individua il tipo ed il numero delle risorse ritenuti necessari a garantire il rispetto degli obblighi connessi alla fornitura del servizio universale assicurando, nel contempo, una gestione economica equilibrata. Ai sensi della vigente normativa, al Ministero delle comunicazioni, quale Autorità di regolamentazione del settore postale, spetta il compito di vigilare affinché i predetti obblighi del servizio universale siano rispettati. Nel passato tale attività è stata prevalentemente finalizzata ad accertare che la qualità del servizio erogato dalle Poste fosse rispondente ai parametri previsti nel contratto di programma che, in particolare, stabiliva gli obiettivi del recapito del corriere postale e a tale proposito le verifiche effettuate hanno consentito di accertare in modo puntuale il raggiungimento o meno degli *standard* fissati. Una parallela efficace azione di controllo relativamente all'accesso alla rete postale non è stata possibile, stante l'indeterminatezza del criterio stabilito in proposito sia a livello comunitario sia a livello di normativa nazionale di recepimento. L'obbligo di fornire il servizio universale «in tutti i punti del territorio secondo criteri di ragionevolezza» (articolo 3 del decreto legislativo infatti, pur con l'individuazione delle «particolari situazioni delle isole minori e delle zone rurali e montane», di cui al decreto legislativo n. 384 del 2003, si è dimostrato non idoneo a consentire una oggettiva valutazione della diffusione e della razionale localizzazione sul territorio nazionale dei punti di accesso alla rete postale e, in particolare, degli uffici postali. Per il superamento della questione posta, con il nuovo contratto di programma per il triennio 2006-2008, in corso di approvazione, si intende garantire l'efficienza del servizio postale senza, tuttavia, intaccare la capillarità della rete soprattutto nei centri più piccoli e nelle aree geograficamente svantaggiate. In particolare, lo schema di contratto di programma prevede che siano individuati - nel periodo di vigenza dello stesso - d'intesa con la società e sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, i parametri relativi alla distribuzione degli uffici postali o dei servizi sul territorio, l'orario di apertura degli sportelli in relazione alle prestazioni richieste e ai tempi di erogazione del servizio, in coerenza con gli impegni assunti dalla società Poste nella Carta della qualità. Ulteriore impegno previsto da parte della società Poste è quello di non dare corso ad interventi di chiusura o di rimodulazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici postali che non siano stati preventivamente comunicati all'Autorità. Quanto al problema dell'orario di apertura va, tuttavia, sottolineato che il decreto legislativo n. 261 del 1999, che regola attualmente l'attività del fornitore del servizio universale, non prevede obblighi specifici al riguardo. La determinazione degli orari rientra, infatti, fra le modalità organizzative lasciate alla libera scelta aziendale, con il solo impegno di rispettare gli obblighi del servizio universale, come, peraltro, precisato anche dal Consiglio di Stato (parere n. 1027 del 2002) che ha riconosciuto a Poste italiane la discrezionalità e l'indipendenza proprie dell'attività di impresa, sotto tale profilo. Nel rispetto di tale autonomia, il Ministero auspica il raggiungimento, a livello locale, di accordi e di intese volte ad evitare la chiusura di uffici postali e ad assicurare un livello soddisfacente di servizi postali anche nei piccoli Comuni, pure se ciò comporta, in alcuni casi, una rimodulazione degli orari di apertura al pubblico. Venendo al problema posto nell'atto ispettivo in esame, la società Poste ha anzitutto precisato di non aver attuato alcun «nuovo progetto *external*» e che, comunque, la trasformazione degli uffici in «*external*» - o «modulari», secondo una nuova definizione - che in Toscana, durante il 2006, ha riguardato solo sei uffici, uffici, non determina variazione nell'orario di apertura, in quanto è riferita alle caratteristiche del collegamento informatico *server*-clienti. II processo che, al contrario, può comportare la variazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici è la riorganizzazione del servizio di recapito in atto su tutto il territorio nazionale, connessa con il superamento della figura dell'operatore polivalente, ossia dell'addetto che nell'arco della giornata lavorativa svolge sia mansioni di sportelleria sia di recapito, in linea con l'obiettivo di calibrare l'offerta dei servizi alla domanda locale, anche in adesione al protocollo di intesa Poste italiane - ANCI Nell'ambito di siffatto generale processo di riorganizzazione aziendale, la società Poste ha previsto una diversa articolazione dell'orario di apertura degli uffici correlata ai reali volumi di traffico registrati nelle singole situazioni locali, per cui può verificarsi che alcune sedi rimangano aperte *full time* limitatamente ad alcuni giorni delle settimana, pur mantenendo e, talvolta, aumentando il numero delle ore settimanali di apertura. Nella Regione Toscana gli interventi di questo tipo hanno interessato 75 uffici, determinando per 41 di essi un aumento complessivo dell'orario di apertura al pubblico, per 21 il mantenimento dell'orario complessivo precedente e per 11 una diminuzione dell'offerta. Solo in 2 casi si è fatto ricorso alla chiusura di uffici, ossia nei casi di Travale e Lago Boracifera, nel Comune di Monterotondo, entrambi situati nella Provincia di Grosseto e rientranti nel piano di chiusure previsto per il 2005, essendo inclusi nell'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, presentato dalla società Poste ai sensi del contratto di programma 2003-2005 (articolo 6, In particolare, nessun ufficio della Provincia di Firenze è stato inserito nella riorganizzazione in parola, mentre in alcuni uffici delle Province di Pisa, Grosseto

Nella Provincia di Massa Carrara, nella Comunità montana della Lunigiana, gli interventi di cui trattasi hanno interessato solo 10 dei 45 uffici ubicati nei 14 Comuni di cui la stessa Provincia si compone. Poste italiane ha, infine, fatto presente che negli ultimi tre anni, grazie al processo di allineamento dell'offerta e alla domanda locale di servizi, è stato possibile attivare 6 uffici *retail* in zone ad alta densità di clientela che ne erano prive, 4 uffici *business* in zone con rilevante presenza di aziende, nonché potenziare gli sportelli negli uffici di maggiori dimensioni, specializzando 67 sportelli dedicati alle aziende e prolungando l'orario di apertura pomeridiana in 4 uffici.

che va nella direzione della sostenibilità della presenza sul territorio degli uffici postali.

delle gestioni contabili dei piccoli uffici postali, una strategia di razionalizzazione e di contenimento dei costi. Il fatto che si sia adottata una strategia esclusivamente di riduzione dei costi fa di questo progetto un qualcosa che indebolisce fortemente la componente sociale del servizio postale universale. Ora, non può sfuggire a nessuno, invece, la rilevanza sociale e culturale della presenza di tali uffici

La Regione Toscana si è fatta carico di alcune proposte estremamente importanti e concrete. La prima, rivolta al Governo e di cui lei stamattina ci ha dato conferma, è che nel nuovo contratto nazionale si riveda al meglio la presenza sul territorio degli uffici postali, eventualmente inserendo preciseclausole sociali per favorire accordi con Comuni, Province, Comunità montane e con le stesse Regioni. In secondo prevedere uffici polifunzionali. E' una novità di cui la Toscana si sta facendo carico perché detti uffici consentirebbero alle Poste di erogare servizi

realizzerebbe attraverso un processo di concertazione, stipulando poi convenzioni in modo tale che gli uffici postali, offrendo questi servizi aggiuntivi, possano avere anche vantaggi economici, il che risolverebbe un importante punto che è alla base del processo di razionalizzazione.

Giusta, quindi, la sensibilità da lei mostrata a nome del Governo, giusto aiutare i territori montani, collinari e svantaggiati, giusto e importante - e lo porto a sua conoscenza e a

salute*. Signor Presidente, per la terapia della sclerosi laterale amiotrofica (SLA), malattia neurodegenerativa progressiva rara, che colpisce in Italia circa 1.500 persone, al momento non esiste un farmaco in grado di curarla o di modificarne il decorso in maniera clinicamente significativa per i pazienti. Il Rilutek (principio attivo riluzolo) è l'unico farmaco dotato di indicazione registrata nell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America per la SLA e costituisce la sola terapia farmacologia che ha mostrato, finora, all'interno di sperimentazioni cliniche, un prolungamento della sopravvivenza di circa tre mesi dei pazienti affetti dalla malattia rispetto al placebo. Il farmaco è indicato nei pazienti con SLA definita o probabile, secondo i criteri della *World Federation of Neurology*, con sintomi presenti da meno di cinque anni, non tracheostomizzati e con capacità vitale forzata maggiore del 60 Attualmente sono oggetto di sperimentazione numerose altre molecole. Recentemente la Società scientifica neurologica statunitense, l'*American Academy of Neurology*, ha pubblicato sulla rivista «Neurology» i risultati di una valutazione rigorosa della letteratura scientifica disponibile sugli agenti neuroprotettori potenzialmente utili nella SLA, allo scopo di identificare quali tra queste molecole meriterebbero di essere prioritariamente studiate nell'ambito di sperimentazioni cliniche di fase (pubblicazione del 2006). In base alle informazioni riportate in questo articolo e a quanto è disponibile nel sito «clinicaltrials.gov», che riporta le sperimentazioni attualmente in corso, è possibile individuare un elenco di circa 20 sostanze che sono al momento nella fase II e III della sperimentazione clinica riguardante la SLA. Tra le molecole di questo elenco, per le quali la necessità di ulteriori sperimentazioni è giustificata dall'assenza di prove di efficacia, è annoverata anche l'IGF-1. Diverse sperimentazioni con altri prodotti sono in corso anche in Italia: due sono state approvate e finanziate dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) all'interno dei bandi di ricerca *non-profit* del 2005 e altri progetti sono in corso di valutazione nei bandi AIFA per il 2006. Per quanto riguarda l'*Insuline-line Growth Factor-*1 (IGF-1), è opportuno ricordare che tale farmaco non è approvato per il trattamento della SLA in alcun Paese del mondo. È stato registrato alla fine del 2005 dalla *Food and Drug Administration* (FDA), per la seguente indicazione: «Trattamento del malaccrescimento in bambini con severa e primaria deficienza di IGF-1 o che presentino delezione del gene GH (ormone della crescita) e che abbiano sviluppato anticorpi neutralizzanti l'ormone della crescita». La ragione per la quale l'IGF-1 non presenta un'indicazione approvata per la SLA, né in Italia né in alcun altro Paese del mondo, dipende dal fatto che le due sperimentazioni finora condotte non hanno mostrato un guadagno clinicamente rilevante per i pazienti. Infatti, i risultati dei due studi sono stati contraddittori: il primo, condotto negli Stati Uniti, ha dimostrato che l'IGF-1 era in grado di migliorare alcuni parametri funzionali dei malati, mentre il secondo, condotto in Europa, non ha fornito prove di superiorità dell'IGF-1 rispetto al placebo. Attualmente è in corso un altro studio americano, che ha coinvolto circa 300 pazienti, i cui risultati dovrebbero essere disponibili forse tra un anno. Nessuno studio ha quindi finora dimostrato che l'IGF-1 sia in grado di migliorare la sopravvivenza o la qualità di vita dei pazienti con SLA: d'altro canto, lo studio americano in corso sottolinea l'interesse da parte della comunità scientifica nei confronti di nuovi trattamenti per la SLA, confermandone tuttavia la natura «sperimentale» e «*in progress*». L'IGF-1/BP3 complex (o mecasermina), segnalato nell'interrogazione, è un composto con proprietà simili all'IGF-1, potenzialmente in grado di rallentare la degenerazione del tessuto molecolare: questo farmaco, tuttavia, non è ancora stato studiato nei pazienti affetti da SLA e, a questo proposito, bisogna evidenziare che, solo all'interno di un contesto di ricerca e di sperimentazione clinica, potrà essere possibile individuare farmaci potenzialmente efficaci nel trattamento della SLA. Inoltre, non può non essere ribadito che la somministrazione di farmaci, il cui profilo beneficio-rischio non venga adeguatamente studiato, espone i pazienti a rischi inutili e non consente di acquisire alcuna informazione valida che sia estrapolabile a vantaggio di tutti gli altri pazienti. Relativamente alla questione dell'erogazione ad uso compassionevole del farmaco IGF-1 per la cura della SLA, si precisa che nel 2002 il tribunale civile di Lamezia Terme (Catanzaro), con ordinanza d'urgenza del 12 febbraio, ordinava al Ministero della salute l'erogazione del medicinale in favore del paziente ricorrente per il tempo necessario alla cura. Presupposto della decisione giudiziale era il protocollo d'intesa siglato dal Ministero il 19 luglio 2001 con le ditte Chiron e Pharmacia, al fine di garantire la somministrazione del farmaco ad uso compassionevole e in base al quale tali aziende si impegnavano ad assicurare, nei limiti della disponibilità, la fornitura del medicinale IGF-1 previa segnalazione del Ministero. Attualmente, secondo quanto comunicato dalle ditte firmatarie dell'accordo, le scorte del farmaco in questione sono completamente esaurite; pertanto, il citato protocollo è ormai senza effetto, come riconosciuto di recente dal tribunale di Siena (ordinanza collegiale del 25 agosto 2006). Esiste peraltro un contrasto interpretativo tra i giudici di merito: a fronte delle ordinanze favorevoli alla fornitura del farmaco, ve ne sono sei contrarie. In particolare, il tribunale di Sassari, sulla base della perizia d'ufficio, ha ritenuto non dimostrate l'efficacia terapeutica del farmaco e la sua insostituibilità per la cura della patologia SLA. Soltanto ove tale possibilità fosse riconosciuta praticabile, infatti, sarebbe possibile l'erogazione gratuita del farmaco; come affermato dalla Corte di Cassazione, «il diritto alla somministrazione di farmaci è attribuito agli utenti del SSN dall'art. 8 della legge n. 537 del 1993, commi 9° e ss., con la mediazione del provvedimento, a carattere generale e conformativo - espressione di discrezionalità amministrativa e non meramente tecnica, considerata la valutazione del rapporto costi-benefici demandata all'amministrazione dell'organo collegiale del Ministero della sanità denominato "Commissione unica del farmaco", competente alla formulazione del giudizio circa il carattere essenziale di un farmaco o la sua significativa efficacia terapeutica ai fini dell'inserimento nelle classi a) o classi a) o b)». Si segnala che la procedura per l'utilizzo del fondo nazionale per l'impiego, a carico del Servizio sanitario nazionale, di farmaci orfani per malattie rare è stata formalizzata in un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA nel maggio 2005. Tale procedura prevede, in particolare, una istanza del richiedente, sulla quale si pronuncia la Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA (CTS): la valutazione tecnica della CTS è necessaria e imprescindibile, al fine di appurare il valore terapeutico dei farmaci, anche con riguardo a quelli che rappresentano una speranza di cura per le patologie rare, e di stabilire la loro possibile somministrazione a carico del Servizio sanitario nazionale. Nei casi di richieste di accesso al fondo, la CTS si pronuncia in ordine alla validità del protocollo di cura presentato, con particolare riguardo all'efficacia rispetto alla patologia per cui viene prescritto. La CTS, nell'approfondire la questione scientifica dell'efficacia terapeutica dell'IGF-1/IGF-1BP3 per la cura della SLA, ha ritenuto che non siano presenti i requisiti minimi per fornire gratuitamente il farmaco IGF-1 a pazienti affetti da SLA; non è, inoltre, da sottovalutare che le rilevanti risorse necessarie per questa terapia (circa 140.000 euro per paziente ogni anno) devono intendersi come sottratte a quei trattamenti terapeutici in possesso di evidenze scientifiche comprovate. Una conclusione simile riguarda anche il farmaco IGF-1/BP3: questo, infatti, è attualmente indicato per il trattamento a lungo termine del *deficit* di crescita in bambini con carenza primaria di IGF-1 o di GH. Si ritiene opportuno, in questa sede, riportare le conclusioni formulate dalla CTS: non vi sono i presupposti per fornire gratuitamente, a carico del Servizio sanitario nazionale (nell'ambito della legge 23 dicembre 1996, n. 648), i farmaci IGF-1 e IGF-1/BP3 per il trattamento di pazienti affetti da SLA; l'utilizzo di IGF-1 e di IGF-1/BP3 nella SLA non è supportato né da strumenti normativi (essendo un farmaco sprovvisto di indicazioni registrate), ne' da evidenze scientifiche (dagli studi conclusi finora non esistono prove che l'IGF-1 sia efficace nella terapia della SLA, mentre l'IGF-1/BP3 non è ancora stato studiato nei pazienti affetti da tale patologia); non sono mai stati indagati esiti rilevanti per il paziente, come la sopravvivenza, quindi in questo senso l'IGF-1 non è un farmaco «salvavita», come talvolta viene definito impropriamente dai mezzi di informazione; le attuali conoscenze scientifiche non giustificano un uso dei prodotti IGF-1 e IGF-1/BP3, al di fuori di una condizione di ricerca. La CTS, peraltro, ritiene che, con una intesa tra il Ministero della Salute, l'AIFA e l'Istituto Superiore di Sanità, possa essere istituito un Tavolo scientifico che dia avvio ad uno studio clinico che verifichi la complessiva efficacia del principio attivo IGF-1 e il suo profilo di beneficio-rischio nei pazienti affetti da SLA, rendendo così valutabile il confronto con il trattamento farmacologico a base di Rilutek, oggi disponibile e a carico del Servizio sanitario nazionale. Per completezza, me lo consentite, vorrei inoltre segnalare che recentissimamente il nostro Ministero ha insediato una Commissione per lo studio della sclerosi laterale amiotrofica e ha stabilito questo accordo insieme all'AIFA per dar vita ad un protocollo sperimentale su tali farmaci.

detto. Sono molto felice che il Ministero abbia messo al lavoro una Commissione per valutare i farmaci e le terapie nei confronti di questa malattia rara,

di una malattia che è importante, che è vero che è rara, ma riguarda molte persone nel nostro Paese e, anche se ne riguardasse una, ce ne dovremmo far carico. Le cose che lei ha detto sono in palese, patente, totale contraddizione con quanto affermato dal Ministro *pro tempore* della XIII legislatura sull'efficacia dell'IGF-1 nell'ottenimento dei risultati brillanti nella cura della SLA, proprio alla luce di dati emersi dalla sperimentazione negli USA.

epidemiologico caso controllo sui sarcomi dei tessuti molli, condotto dall'Istituto superiore di sanità per approfondire le segnalazioni dell'Istituto tumori di Milano, ha indotto l'ASL di Mantova ad istituire una commissione di studio coordinata dal dottor Ricci, all'epoca direttore del dipartimento di prevenzione dell'azienda, e della quale facevano parte il dottor Pietro Comba ed il dottor Lorenzo Tomatis. cercherò di essere meno freddo e più partecipe nella risposta. Spero quindi di accontentarla. La commissione, che si è avvalsa della collaborazione del laboratorio di riferimento mondiale "CDC" di Atlanta, ha prodotto, nell'ambito del «Piano di monitoraggio ambientale ed epidemiologico per gli specifici inquinanti associati alle produzioni industriali del polo chimico di Mantova» realizzato dalla ASL mantovana, lo «Studio della concentrazione di diossina nel sangue di due campioni di popolazione mantovana a diversa incidenza di sarcoma dei tessuti molli», il quale ha esaminato la concentrazione di diossina nel sangue in un campione della popolazione mantovana, comprendente soggetti residenti sia nella zona immediatamente circostante l'area industriale sia nel centro storico. La ricerca ha evidenziato un'alta concentrazione di Odds Ratio, calcolata per tali sarcomi, nel sangue delle persone con dimora nella città, a prescindere dal fatto che esse risiedessero nella zona più limitrofa agli impianti industriali o vivessero oltre il raggio di due chilometri dal polo chimico cittadino. L'esito descritto non ha mancato di determinare un forte allarme nella popolazione, anche in considerazione dell'elevata presenza di diossina che sembrerebbe essere stata riscontrata nel sangue delle persone esaminate e che avrebbe raggiunto picchi superiori al doppio del limite di tolleranza. Relativamente all'avvenuto avvicendamento alla guida dell'*équipe* di ricerca incaricata dello studio in esame, voluto dal direttore generale *pro tempore* della ASL, nonostante le richieste, non sono pervenute al Ministero precisazioni in merito; tuttavia, l'attuale responsabile dell'azienda ha ribadito il costante impegno affinché tra il gruppo di ricerca originario e la nuova *équipe* medica possa realizzarsi la più proficua collaborazione, precisando che al dottor Ricci è stato attribuito l'incarico di responsabile dell'Osservatorio epidemiologico della ASL di Mantova, a riconoscimento delle sue capacità professionali e della preparazione scientifica. Per quanto di competenza di questo Ministero, si precisa che con decreto ministeriale del 31 agosto 2000 era stata istituita una commissione nazionale «per lo studio della situazione igienico-ambientale in relazione al polo chimico di Mantova e per la individuazione di proposte operative di intervento». La commissione ha concluso i propri lavori nel marzo 2003, producendo un rapporto conclusivo che suggeriva l'esecuzione di una serie di ulteriori analisi di approfondimento da parte della competente azienda sanitaria. La stessa azienda successivamente ha fatto pervenire al Ministero uno «Studio della concentrazione ematica di diossine, furani e PCB in due campioni della popolazione di Mantova», conclusosi il 20 luglio 2006; dei risultati di tale studio è stata data notizia con il comunicato stampa di questa Amministrazione del 1° agosto 2006. Occorre precisare che lo studio, realizzato dal Professor Bertazzi della Clinica del lavoro «Luigi Devoto» dell'Università degli studi di Milano, ha sottolineato che «complessivamente, i risultati di questa indagine non hanno messo in luce differenze di rilievo nei livelli plasmatici di diossine, furani e PCB tra residenti vicino al petrolchimico e residenti nella zona centrale della città di Mantova». Le risultanze sono state fatte proprie dalle autorità sanitarie regionali a cui era stata attribuita la supervisione dello studio, con la raccomandazione di continuare l'indagine attraverso la valutazione della contaminazione di vegetali, latte ed altre matrici ambientali nelle aree del polo chimico di Mantova. Nell'ambito del citato progetto Piano di monitoraggio ambientale ed epidemiologico veniva realizzata un'ulteriore indagine rivolta alla misurazione dei livelli ematici di varie sostanze diossino-simili (*dioxin-like*), in un gruppo di soggetti residenti in zona industriale ed in un gruppo di soggetti residenti in centro città. Questa iniziativa era finalizzata ad approfondire, dietro suggerimento della commissione istituita dall'ASL di Mantova, le analisi dei dati che nella precedente relazione mostravano la presenza di livelli di alcune sostanze lievemente più elevati nella zona industriale rispetto al centro cittadino, nonché a realizzare una sintesi dei risultati della rassegna bibliografica sui livelli ematici di equivalenza tossica (TEQ), in campioni di popolazione non professionalmente esposta e residente in zone considerate non contaminate. I risultati di tale monitoraggio biologico sono stati presentati il 1° dicembre 2006 a Mantova, nell'ambito del convegno «Diossina e rischio per la salute». Complessivamente, tali risultati hanno messo in luce moderate differenze nei livelli plasmatici di alcuni furani e bifenili policlorurati (PCB) tra i residenti vicino al petrolchimico e i residenti nella zona centrale della città di Mantova: un eventuale ruolo di tale moderato incremento nel causare il forte eccesso di STM riscontrato nell'area. Dalla rassegna bibliografica è emerso, altresì, che i valori determinati nella popolazione di Mantova, pur collocandosi su valori medio-alti per tutti i tipi di TEQ, sono all'interno dell'arco di valori misurati in numerosi altri studi in popolazioni non esposte; tale affermazione risulta rafforzata dal fatto che l'età dei soggetti di Mantova (69-70 anni) era molto superiore a quella presa in considerazione da altri studi (persone meno di 50 anni). 50 anni). Pertanto, si può affermare che i valori di TEQ riscontrati nei campioni della popolazione di Mantova rientrano nell'arco di quelli usualmente misurati nella popolazione generale non esposta professionalmente e residente in aree non contaminate. Peraltro, il Ministero della salute, allo scopo di garantire maggiore informazione alla popolazione interessata e soprattutto il monitoraggio della situazione di rischio per la salute, auspica, in accordo e nel rispetto delle autorità locali, l'istituzione di un tavolo tecnico permanente, con la presenza di tutti gli esperti interessati da tempo a tale problematica. Si segnala, infine, che l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ha affidato al Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute il compito di acquisire e certificare i Piani regionali di prevenzione 2005-2007; per l'anno 2005 il CCM ha stabilito che le Regioni sono tenute a presentare i Piani regionali relativi alla prima fase delle linee operative, tra i quali anche quelle riguardanti gli *screening* oncologici. Tutte le Regioni e Province autonome hanno predisposto i progetti esecutivi e i relativi cronoprogrammi (strumenti per verificare lo stato di avanzamento di ciascun progetto, la relativa attuazione ed il suo discostarsi dalle previsioni, anche al fine di poterlo modificare e migliorarlo in *itinere*), ottenendo la certificazione da parte del CCM. Gli Enti regionali hanno avviato, altresì, la fase di realizzazione dei programmi di prevenzione già certificati dal CCM. Per quanto riguarda, in particolare, la Regione Lombardia, si precisa che la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. VIII/00217 del 27 giugno 2005, la prima parte delle linee operative del Piano regionale di prevenzione attiva 2005-2007, il quale delinea, tra gli altri, anche con i seguenti progetti: *screening* del carcinoma della mammella nella Regione Lombardia; progetto di attivazione di un programma di *screening* del carcinoma colon rettale mediante ricerca di sangue occulto fecale. Con la stessa deliberazione sono stati quantificati in via previsionale stanziamenti pari a 40.000.000 euro per interventi di *screening* oncologici, da avviare entro il

credo che non dovrei essere io a dichiararmi non soddisfatto da questa risposta ma dovrebbe essere il Governo a dichiararsi non soddisfatto della risposta che è stata presentata dagli uffici soprattutto delle mancate risposte a livello locale, cosa direi piuttosto grave, anche perché sono state fornite delle indicazioni, perfino da un punto di vista scientifico e di accertamento specifico assolutamente non corrette e non corrispondenti ai documenti. Nei pochi minuti che ho non posso certamente affrontare nel dettaglio questa situazione. Cercherò però di dare alcune indicazioni, proprio per vedere se è possibile che il Governo si interessi maggiormente a questa situazione, anche al di là di una sollecitazione da parte del Senato. Qui avevamo un dato di partenza che risale al 1996-97, pubblicato nel primo numero della rivista «Epidemiologia e prevenzione» del 1998, in cui veniva segnalata l'anomala presenza di sarcomi dei tessuti molli, in particolare nella zona industriale di Mantova.

veniva indicato che vi era un eccesso proprio dei sarcomi dei tessuti molli e veniva confermata l'associazione tra tale sarcoma e la distanza della residenza rispetto all'inceneritore, con un indicazione numerica di 31,4 rispetto a un valore atteso di uno, quindi l'indicazione era estremamente forte. È stato dato incarico ad un centro internazionale di Atlanta negli Stati Uniti, proprio per confermare questi dati; erano stati coinvolti l'ex direttore dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, professor Tomatis, e l'Istituto superiore di sanità. Questi dati, nella sostanza, venivano confermati. A un certo punto, in maniera incomprensibile, vi è una sostituzione di questi esperti di fama e di capacità mondiale con interventi di altre persone e di altre cliniche,

proprio secondo quella che era l'ottica iniziale: una associazione tra esposti in zona industriale e aumento dei sarcomi nei tessuti molli.

Ancora più interessante è rilevare come in queste conclusioni del dicembre 2006 la clinica Devoto di Milano segnalava: "Rimane da discutere la rilevanza del dato nello spiegare l'aumento di questi sarcomi". Ora, dal 1996 sono passati dieci anni

un rapporto della Commissione Europea dell'ottobre del 1999 in cui si parla espressamente di riduzione, per quanto possibile, delle diossine nell'ambiente, di identificazione dei gruppi maggiormente esposti e a rischio di danno da contaminazione da diossina e di raccomandazione relativamente all'esposizione per via alimentare. la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale in materia di diossine, furani e bifenili policlorurati è dello stesso tenore. Ora, per questo, signor Sottosegretario, mi permetto di insistere, proprio per valutare se non sia veramente il caso,

che superano grandemente la media generale italiana e anche di altre zone industriali, non solo europee, ma del mondo.

utilizzato per il reinventario dei beni mobili di tutte le Amministrazioni dello Stato, le cui scritture contabili devono essere gestite con modalità informatiche. Al riguardo, sentito il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si fa presente che il nuovo Sistema di Gestione e Controllo dei beni mobili dell'Amministrazione statale (GECO), di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze, è un'evoluzione dell'applicazione Funzioni Locali degli Uffici (cosiddetta FLU), già in uso presso le Ragionerie provinciali dello Stato dal 1997 e diffusa nell'anno 2001 ai Dipartimenti provinciali, per assolvere alle operazioni di rilevazione, riscontro e controllo della gestione dei beni mobili in loro dotazione. A seguito dell'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, recata dal decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e del successivo riassetto organizzativo dei Dipartimenti del neocostituito Ministero, avviato con decreto ministeriale 8 giugno 1999, il Provveditorato generale dello Stato è stato soppresso. Inoltre, con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, è stata attribuita a questo Ministero la competenza sulle attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile; tale competenza, con decreto del 22 dicembre 1997, è stata affidata alla propria partecipata Consip S.p.a (il 100 per cento del capitale sociale della quale è detenuto dal Ministero). L'esigenza di rivedere le procedure informatiche relative alle Funzioni Locali degli Uffici (ex FLU), in ordine alle scritture contabili dei consegnatari, è scaturita dalla rivisitazione della normativa, a partire dal 2002: Repubblica n. 254 del 2002, concernente il regolamento delle gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 aprile 2002, riguardante la nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato, il cosiddetto SEC 95, al quale sono seguite le circolari applicative n. 2 del 16 gennaio 2003 e n. 13 del 12 febbraio 2003. Conseguentemente, questo Ministero, alla luce delle competenze derivanti dal citato decreto in materia informatica, finanziaria e contabile, ha ritenuto opportuno, con la circolare n. 41 del 15 novembre 2002, estendere alle Amministrazioni statali la possibilità di utilizzare il prodotto GECO, previa adesione volontaria e gratuita (lo sottolineo: volontaria e gratuita). L'applicativo consente un più agevolato svolgimento dei compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica affidati agli Uffici di Ragioneria provinciali ed agli Uffici centrali di Bilancio, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il sistema GECO si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: possibilità di avere, a livello centrale ed in tempo reale, informazioni dettagliate sulla consistenza e sulla ripartizione del patrimonio dello Stato; maggiore velocità e precisione del controllo effettuato dagli Uffici di Ragioneria sulle gestioni dei consegnatari ad essi sottoposti; eliminazione di tutti i modelli cartacei; integrazione automatica con il Sistema Informativo Patrimonio e con i sistemi conoscitivi di pertinenza della Ragioneria Generale dello Stato; produzione di statistiche ed analisi sulla ripartizione della spesa in beni mobili tra uffici centrali e periferici dell'Amministrazione; economie di bilancio sempre maggiori, in conseguenza dell'utilizzo di un'unica procedura *standard* per tutte le Amministrazioni statali, garantendo, tra l'altro, la sicurezza dei dati nazionali. La recente introduzione dei concetti di ammortamento e di contabilità economica per centro di costo, nonché il rinnovo inventariale, di cui alla circolare n. 42 del 2004, hanno reso necessario un aggiornamento della procedura (GECO 2), realizzato con la collaborazione della società Consip nel rispetto della legislazione vigente. Nell'intento di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione, l'articolo 1, comma 192, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), ha promosso la diffusione del sistema attraverso la pubblicazione nel catalogo del riuso *software* del CNIPA, consentendone, così, l'utilizzo da parte di altre pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'applicativo GECO, ha inteso offrire gratuitamente un servizio che agevola la gestione dei consegnatari e i compiti degli uffici di Ragioneria, consente il monitoraggio della spesa e garantisce un aggiornamento ed una formazione professionale degli addetti, offrendo al suo interno un corso di autoistruzione, nonché una raccolta di tutte le norme e circolari in materia. Per quanto concerne, poi, il quesito relativo ai costi, si fa presente che il prodotto attualmente in uso ha comportato un onere globale per il bilancio dello Stato pari a 160.000 euro. Considerato che a tutt'oggi gli uffici che hanno aderito al servizio sono oltre 2.500 e che i consegnatari dell'Amministrazione statale sono 7.200, un utilizzo totale di tale procedura consentirebbe, rimanendo invariato il costo complessivo, un notevole risparmio per il bilancio dello Stato;

Grazie

mi riservo di dimostrarle che le amministrazioni dello Stato, nell'aderire al sistema GECO, hanno dismesso e disdettato i contratti precedenti con gli amministratori privati, facendo riferimento ad un obbligo che sarebbe stato loro imposto da precise disposizioni del Ministero. Non ho potuto

documenti in mio possesso, infatti, risulta che i sistemi utilizzati in precedenza,